Comunico che in data 7 luglio 2010 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo» colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente. La commemorazione dell'ex senatore Pietro Milio, già prevista per questa mattina, avrà luogo martedì 13 luglio, alle ore 11; quella dell'ex senatrice Rina Gagliardi in apertura della seduta pomeridiana di giovedì 15 luglio; quella dell'ex senatore Egidio Sterpa in apertura della seduta pomeridiana di martedì 20 luglio. In relazione alla richiesta unanime della 5a Commissione permanente di poter disporre di ulteriore tempo per concludere l'esame del decreto-legge sulla manovra economica, le sedute già previste per il pomeriggio di oggi e domani mattina non avranno luogo. la discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea avrà inizio nella seduta antimeridiana di martedì 13 luglio e proseguirà nel pomeriggio dello stesso giorno, nonché nelle due sedute di mercoledì 14, per concludersi nella seduta antimeridiana di giovedì 15 luglio. Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea è stabilito per le ore 17 di lunedì prossimo. Si ricorda la convocazione del Parlamento in seduta comune oggi,

a conclusione del decreto-legge sulla manovra economica, quindi a partire dalla giornata di giovedì 15 luglio, sarà esaminato il decreto-legge in materia ambientale e di autotrasporto, già approvato dalla Camera dei deputati.

come tutti ricordano, nello scandalo del G8: scandalo che ha generato un vero e proprio terremoto e ha coinvolto alcuni personaggi eccellenti

Per noi, per l'Italia dei Valori, è una vergogna che deve finire.

Da quella inchiesta giornalistica di altissimo livello è emerso che due degli assassini di Angelo Mancia, militante di destra ucciso il 12 marzo 1980 nel quartiere Talenti,

interverrà per sollecitare la risposta a questa interrogazione con le motivazioni di urgenza e di serietà con cui anche lei ha sottolineato tale richiesta. **Mozioni,